posso riferire che il caso riguarda un detenuto di media sicurezza ristretto presso la casa circondariale di Torino il quale, dopo essere stato allocato presso il padiglione soggetti a riprovazione sociale e a trattamento intensificato, è stato assegnato al padiglione A sezione SAI, che sarebbe il Servizio di assistenza intensificata, e successivamente trasferito presso la sezione circondariale infermeria annessa al SAI in ragione delle sue delicate condizioni di salute. Considerate le ragioni per le quali il ristretto ha iniziato lo sciopero della fame e della sete, l'amministrazione si è già da tempo attivata trasmettendo una nota interlocutoria all'ufficio competente presso la Repubblica di Albania in mancanza di riscontro, si è di recente altresì provveduto ad inviare un nuovo sollecito. Del caso si è interessato anche il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per il Piemonte, il quale ha inviato una lettera al Consolato generale della Repubblica di Albania, con cui ha comunicato che l'interessato era in sciopero della fame e manifestava la ferma volontà di espiare la propria pena nel Paese di origine, subendo perciò un ricovero e rifiutando ogni trattamento a tutela della sua salute. Quanto alla gestione dell'emergenza, trattandosi di soggetto non nuovo a simili proteste, il caso veniva seguito con grande attenzione sia dalla direzione penitenziaria che dalla locale ASL. La direzione penitenziaria ha adottato tutti i necessari interventi per dissuadere il detenuto dal proseguire lo sciopero della fame, predisponendo ogni misura trattamentale e di vigilanza atta a impedire comportamenti autolesionistici, attivando lo specialista psichiatra e aggiornando costantemente la competente autorità giudiziaria, il provveditorato regionale di Torino e la stessa amministrazione. L'area trattamentale, per quanto di sua competenza, ha intensificato i colloqui con il detenuto e ha attivato i gruppi di attenzione per il prosieguo della presa in carico psicologica. Il 21 febbraio scorso la direzione ha comunicato al Dicastero che il ristretto, nel frattempo rientrato in istituto a seguito della dimissione dal reparto detentivo ospedaliero, aveva interrotto l'astensione dall'assunzione di cibi solidi e liquidi, riprendendo ad alimentarsi correttamente. L'approccio assunto dall'amministrazione per far fronte alle criticità connesse alla vicenda oggetto dell'interrogazione costituisce prova tangibile della grande attenzione che il Ministero, a mezzo del preposto dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dedica al tema della prevenzione del suicidio, portando avanti molteplici attività e iniziative. A questo proposito, merita attenzione la nota circolare, adottata l'8 agosto del 2022 dal capo del dipartimento, a seguito di una riflessione condivisa con i provveditori e i direttori di istituto del territorio nazionale, in considerazione dell'aumento dei suicidi nell'anno 2022, e questo ovviamente rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Con suddetta nota, è stata ribadita a tutti i provveditori e i direttori di istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate, in particolare dal 2016 in poi, rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute. Al riguardo, si è attivato un percorso nazionale di intervento continuo sul tema attraverso il quale il citato dipartimento, i provveditorati, gli istituti penitenziari sono tutti coinvolti, in una prospettiva di rete necessaria nella prevenzione di tali drammatici eventi. È stata altresì evidenziata l'importanza di instaurare collaborazioni con l'ordine degli avvocati, al fine di stimolare un canale diretto di comunicazione con l'istituto, nel caso emergano situazioni di rischio per le persone detenute, anche sulla base di quanto il difensore abbia appreso dalle famiglie dei detenuti nonché, a livello locale, con la magistratura e con i garanti. Si è sottolineata, anche di recente, la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto essenzialmente dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggiamento, controllo della persona, verifica dell'eventuale disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario penitenziario da parte dei *supporter* per la chiusura della procedura. Inoltre, in data 20 ottobre 2022, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Tra le tante finalità di tale accordo, si prevede di definire un diverso e più strutturato coinvolgimento degli esperti, ex articolo 80 della legge sull'ordinamento penitenziario, nel trattamento, oltre che nell'osservazione e in particolare nella prevenzione del rischio suicidario. Di recente sono state infine avviate delle interlocuzioni, anche con l'ispettore generale dei cappellani penitenziari, per allargare la platea dei soggetti che possono concorrere fattivamente a compiere tutti gli interventi possibili per la prevenzione dei suicidi, coinvolgendo proprio coloro che quotidianamente svolgono la propria missione a contatto con i detenuti e che, grazie alla spiccata sensibilità che connota il loro approccio, sono in grado di cogliere con il dialogo, l'incontro e la preghiera, i segnali di malessere e di disagio dei reclusi, segnalandoli tempestivamente.

molto più alla portata, che sono già state stabilite in un protocollo d'intesa tra i due Paesi per agevolare il trasferimento, qualora venisse richiesto, mi sembra di aver capito che, nonostante

su 1.064 posti regolamentari, abbiamo 1.450 detenuti. È di questa settimana l'ennesimo suicidio nella casa circondariale «Lorusso e Cutugno». Quanto lei ci ha rappresentato, a nome del Ministro e del Governo, sulla questione più specifica delle condizioni psicologiche e psichiatriche, è ancora del tutto generico. I protocolli cui lei ha fatto riferimento cui lei ha fatto riferimento sono delle petizioni di principio. Qui parliamo di numeri, di provvedimenti concreti che non possono che essere adottati e che sono assolutamente alla portata. Parliamo del fatto che ci sono cinque psichiatri addetti all'istituto penitenziario «Lorusso e Cutugno» a fronte di oltre 3.500 prestazioni e del fatto che si continuano a non fare colloqui di primo ingresso con gli psicologi dell'ASL. Se non Se non parlassimo di cose davvero tragiche, drammatiche, proporre un colloquio con il cappellano a persone che sono a rischio di atti anticonservativi e di suicidio mi sembra obiettivamente

personale operante negli istituti penitenziari è ancora in altissimo mare, e non lo diciamo noi, ma lo dicono i sindacati. Ci sono delle carenze di organico assolutamente drammatiche.

18, e stiamo parlando ancora di numeri insufficienti. Quindi, ancora una volta, sul tema delle carceri e dell'espiazione della pena

migliori di quando sono entrate - siamo ancora assolutamente agli annunci, a provvedimenti contraddittori e alla genericità di protocolli che non prevedono neanche interventi concreti.

tutele e prevenzione proprio per il settore specifico dei macchinisti ferroviari. Inoltre, Presidente, colgo l'occasione di questo momento per rendere noto all'Assemblea pochi giorni fa il Comune di Sulmona, la mia terra di origine, è stato selezionato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri all'interno di un ristretto numero di realtà virtuose per quanto riguarda la gestione di progetti finanziati con i fondi del PNRR in ambito di innovazione tecnologica e digitalizzazione.

in particolare al già assessore Attilio D'Andrea che, tra le altre deleghe, ha esercitato proprio quelle sul PNRR, digitalizzazione e transizione ecologica, e si è speso tanto per questo, a dimostrazione del fatto che la buona politica, quella fatta con la testa, con il cuore e soprattutto con